una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, dopo pochi mesi ci troviamo a esaminare una nuova manovra economica. in realtà correggere, dicendo che ci troviamo a ratificare una nuova fiducia al Governo: ancora una volta, infatti, in quest'Aula è approdato un testo blindato e inemendabile, sul quale far calare la scure del voto di fiducia, pratica che verrà espletata nella giornata di oggi. Al di là dell'ironia, vorrei innanzitutto cogliere un problema metodologico. Questo decreto-legge, presentato dal ministro Padoan come una mera correzione tecnica di bilancio richiesta dall'Europa per il valore di 3,4 miliardi di euro, via via una metamorfosi kafkiana. Il testo al nostro esame somiglia più alle leggi finanziarie della prima Repubblica che a un intervento chirurgico correttivo dei conti pubblici. È così elefantiaco e disomogeneo che risulta faticoso perfino tirare le fila del suo contenuto. D'altra parte, signor Presidente, vi è un indicatore

contenuti nel testo e nelle relazioni che lo illustrano abbondano. Infatti, in questo provvedimento partiamo dallo *split payment*.

ma io temo si concretizzerà in una vera e propria tassa sulla liquidità per imprese, professionisti e fornitori di beni e servizi per la pubblica amministrazione. Passiamo poi alla cosiddetta*web* *tax*, che non è una vera e propria tassa, ma piuttosto un concordato che sana il contenzioso tra lo Stato e le multinazionali non hanno versato le dovute imposte al nostro Paese. Si giunge dunque alla tassa sulle locazioni brevi, meglio conosciuta come "tassa

tassa rischia non solo di soffocare uno dei pochi settori - indicato come *sharing economy* - che ancora mostra segni di vitalità nella nostra economia, ma anche di impedire all'Italia di superare l'attuale inadeguatezza ricettiva rispetto alla domanda e agli *standard* internazionali. Ci sono poi gli aumenti di accise - non mancano mai - e le clausole di salvaguardia sull'IVA, rispetto alle quali voglio ricordare, perché credo sia doveroso, che l'ex premier Matteo Renzi, sul finire del suo mandato, ci aveva detto di "stare sereni": ovviamente sono ancora lì, come una mannaia pronta ad abbattersi sui già molto timidi segnali di ripresa dei consumi degli italiani. In sostanza, in questa manovra non c'è un filo conduttore che vada nella direzione dello sviluppo, che resta una parola magica da evocare in *slogan* pubblicitari senza trovare poi attuazione nei testi normativi, tanto meno negli indicatori dell'economia reale. Signori del Governo, dove sono le misure a favore di piccoli imprenditori, liberi professionisti e commercianti? Da quale articolo di questo lungo testo coloro che alzano una saracinesca, aprono un'azienda

negli imprenditori che, tanto per dirne una, stanno ancora aspettando quantomeno il taglio dell'IRES, promesso ormai più di due anni fa? la mancanza di un filo rosso ha anche alcune piccole convenienze. Sulla carta vengono finalmente aboliti gli studi di settore, mostri burocratici che rendevano per i liberi professionisti più conveniente limitare il fatturato anziché farlo crescere. Questo è un fatto positivo,

di affidabilità non si limitino a cambiare nome a una sostanza che non cambia. Il dubbio è legittimo: non vorremmo che, anche in questo caso, spuntasse qualcuno a dirci - e pure questa è storia e va ricordata, per quanto paradossale - «cucù, gli studi di settore non ci sono più», per poi ritrovarci fra qualche mese con amare sorprese. di questo aspetto, in ogni caso, è arduo trovare in questi 67 articoli qualche misura di supporto al tessuto imprenditoriale. Né si può sostenere che lo sviluppo possa passare per una *spending review* di 460 milioni di tagli in capo ai Ministeri. Per tutta una legislatura abbiamo tagliato soprattutto commissari alla *spending review*; ora questa dichiarazione di intenti, non corredata da misure d'implementazione immediata, fa pensare a un intervento più estetico che di sostanza. A meno di un anno dalla fine della legislatura risulta infatti difficile che i Dicasteri italiani dimostrino autonomamente quella capacità di razionalizzazione della spesa quella capacità di razionalizzazione della spesa che non hanno manifestato negli ultimi tre anni. Questo decreto-legge *omnibus* riflette plasticamente, a me pare, le mutevoli esigenze elettorali non tanto del PD, Grazie

se strutturato flessibilmente, in funzione delle peculiarità dei diversi territori, rappresenta l'unica strada seria per responsabilizzare il governo degli enti locali senza attentare alla loro autonomia né tornare a un centralismo che non ha più alcuna possibilità storica di affermarsi. Signori del Governo,

terreno sia stato fatto l'esatto contrario rispetto a ciò che si sarebbe dovuto fare. Se si ritiene che i *voucher* siano uno strumento utile per la regolamentazione di lavori saltuari e occasionali questo è il nostro avviso - li si sarebbe dovuti difendere affrontando la campagna referendaria, perché a volte in politica bisogna avere il coraggio delle proprie idee, anche quando si parte da posizioni svantaggiate. Signor Presidente,

perché era dato per scontato che quel *referendum* sarebbe finito con un'affermazione dei sostenitori della riforma. Le cose si sono invertite, perché in politica gli argomenti - i buoni argomenti - hanno un peso. Non tutto è tattica e non tutto è comunicazione. li si sarebbe dovuti dunque difendere e, per non essere sordi di fronte alle criticità, si sarebbe dovuta proporre una razionalizzazione che rendesse tale strumento più funzionale e ne impedisse un impiego eccessivamente disinvolto. Invece si è scelto di sottrarsi al giudizio dei cittadini e ora, anziché una razionalizzazione, viene proposta una soluzione che appare più complessa e macchinosa della precedente. Una soluzione legittimamente criticata da quanti erano a favore del *referendum* abrogativo, ma comunque al ribasso anche per chi, come noi, si aspettava che questo strumento venisse difeso e reso più efficiente e ora si ritrova con un *surplus* di burocrazia. Qualsiasi compromesso, in questo Paese, viene effettuato aumentando la burocrazia e le difficoltà per i cittadini. E questo è un grande capitolo, che investe la scuola, l'università e l'economia, che dovremmo avere il coraggio di aprire. Infine, mi pare ci sia un assente in questa manovra: il Sud. Dopo la stagione dei patti-*spot*, finiti nel nulla della propaganda prereferendaria, nemmeno in questa sede hanno trovato spazio

che per attrarre capitali produttivi nel Mezzogiorno sia indispensabile trattare con la Commissione europea un piano di fiscalità di vantaggio, che sia realmente efficace, che aiuti il Sud a colmare il divario che unitamente ad altre condizioni di contesto non consente oggi a quest'area del Paese di ripartire. Da indiscrezioni di stampa sembrerebbe che in un separato e successivo decreto, approvato nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, sia stata proposta l'istituzione di zone economiche speciali

Per quanto ci riguarda lo abbiamo proposto da tempo, abbiamo già elaborato una proposta di legge e uno studio di fattibilità anche finanziaria di una misura di questo tipo e, se le indiscrezioni troveranno conferma,

a beneficio delle località colpite dal terremoto del Centro Italia. Anche questa, signori del Governo, era una richiesta che avevamo avanzato con insistenza sin dal primo momento. Avremmo sperato in una battaglia in sede europea per ampliare la portata dell'intervento, ma la direzione intrapresa è quella da noi auspicata. Più in generale, tuttavia, riguardo alle politiche di risposta all'emergenza del terremoto e, soprattutto, della ricostruzione, occorre anche in questa sede sottolineare come le frammentarie misure proposte dai due Governi succedutisi e disseminate in almeno quattro decreti-legge e in altrettanti disegni di legge,

chiederei anche alla Presidenza del Senato di considerare la possibilità di cambiare l'oggetto della Commissione d'inchiesta la cui istituzione è stata approvata, perché oggi una Commissione d'inchiesta sul sisma dell'Aquila, senza che ci sia una comparazione con quello che è stato fatto nei drammi successivi,

La rideterminazione della base ACE, che era un aiuto alla crescita economica, che stava dando qualche piccolo risultato,

Quindi si farà cassa con lo *split payment*, si toglierà liquidità alle aziende

quello che vuol fare, non può lasciare la questione indeterminata e impedire alle Province di fare un minimo di programmazione. Non si può lasciare lasciare che le Province non riescano a svolgere il loro ruolo fondamentale che i cittadini hanno comunque deciso di lasciargli

poi però si è ricordato di aumentare lo stipendio

soprattutto alla fiducia a questo Governo, che assolutamente non la merita. questo decreto-legge, nato con obiettivi di aggiustamento dei conti pubblici da noi condivisi e via via trasformatosi in un decreto *omnibus*, contiene un *vulnus* democratico che non possiamo ignorare. dall'inserimento dei nuovi *voucher* nella manovra, una scelta non accettabile nel metodo, perché si tratta di un aggiramento della domanda referendaria sottoscritta da più di tre milioni di cittadini, e nel merito, perché fallisce l'obiettivo dichiarato di combattere il lavoro nero. È stato il Governo a decidere l'abolizione integrale dei *voucher*, dopo aver perso un anno senza avviare alcun confronto sui quesiti referendari innanzitutto con i promotori (la CGIL). Se si riteneva che i *voucher* andassero diversamente regolati, bisognava allora fare un'altra cosa: adottare una nuova disciplina, non abrogarli, e se questa nuova disciplina non superava le ragioni del *referendum*, bisognava sottoporla al voto dei cittadini. Così facendo, invece, si introduce un precedente grave: la maggioranza di turno potrà sempre neutralizzare un *referendum* non gradito abrogando la norma oggetto del *referendum* per reintrodurla poi, con qualche modifica, qualche giorno dopo. giorno dopo. Non va bene. Soprattutto per una maggioranza che si richiama al centrosinistra. Nel merito, poi, non c'era un vuoto normativo. Per le imprese, in particolare, esiste una pluralità di strumenti contrattuali che assicurano la cosiddetta flessibilità: la somministrazione di lavoro, il lavoro a chiamata, il *part-time*, la surroga e l'extra. L'introduzione di nuovi *voucher* non deriva da una assenza di flessibilità del lavoro, ma dalla volontà di ridurne il costo riducendo tutele e diritti. Per quanto i nuovi *voucher* abbiano un costo superiore ai vecchi e diano una copertura previdenziale più alta, la differenza fondamentale dalle forme contrattuali

ci sono tre giorni per revocare la dichiarazione di utilizzo, ma in assenza di controlli si può dire che la prestazione non ha avuto luogo e pagarla in nero. Altro che lotta al lavoro nero. Questo è il punto. C'è troppa precarietà in giro, soprattutto per i giovani. Non scarseggia solo il lavoro, troppo spesso c'è mancanza di dignità del lavoro. C'è umiliazione. Senza diritti, senza una maggiore stabilità del lavoro non ci sarà una solida ripresa dei consumi, né una crescita vera. Questo strappo poteva e doveva essere evitato. Se proprio si voleva disciplinare nuovamente questa materia, si doveva farlo con misure ragionevoli, a cominciare dal lavoro occasionale per le famiglie, con un provvedimento specifico, rispettoso delle prerogative del Parlamento dopo un confronto con le parti sociali e non con la riformulazione di un emendamento, non subemendabile, in un decreto-legge su cui è stata posta la fiducia sia alla Camera che al Senato. Per questa ragione abbiamo detto: togliete la norma sui *voucher* e votiamo la fiducia. 5a Commissione abbiamo ritirato nostri emendamenti, compreso quello (a cui tenevamo molto) contrario all'ennesimo condono fiscale, lasciando solo quello soppressivo sui *voucher*. Volendo, i tempi tecnici per un ultimo passaggio alla Camera c'erano; il Governo e la maggioranza, invece, hanno tirato diritto insistendo su una scelta divisiva che altri hanno voluto, non noi. Il nostro dissenso sui *voucher* non ci impedisce di vedere alcune cose buone nel decreto-legge in esame: le misure a favore delle aree terremotate, quelle per Comuni e Provincie, sia pure in un quadro ancora precario ed precario ed emergenziale; le misure per il contrasto all'evasione dell'IVA. Non mi riferisco certo al condono mascherato con la rottamazione dei contenziosi, né certo agli 8 milioni dati ad un privato quando tutto il teatro italiano boccheggia. Conosciamo la condizione del Paese: la ripresa economica è ancora insufficiente, esposta ai rischi di nuovi *shock* interni ed esterni. La crescita degli investimenti e il contrasto alle diseguaglianze e alle povertà si devono fare senza sfasciare i conti pubblici si possono finanziare con la riduzione delle spese improduttive, con una distribuzione più equa del prelievo fiscale, con la lotta all'evasione fiscale. Sarebbe bene, quindi, approvare la legge di bilancio prima delle elezioni politiche, senza salti nel buio. In vista di questo appuntamento, la nostra priorità rimane sempre la stessa, cioè affrontare il disagio popolare: investimenti e non sgravi; stop ai *bonus* a pioggia; diritti del lavoro da ricostruire; progressività fiscale, scuola e sanità pubbliche da rilanciare. In altre parole, per noi la prossima legge di bilancio deve contenere novità vere, deve avere cambiamenti reali. Ci sono, poi, altre cose urgenti e rilevanti da fare nei prossimi mesi: la legge sulla cittadinanza e il testamento biologico. Norme di civiltà già approvate dalla Camera che riguardano la vita di centinaia di migliaia di cittadini, che dopo un lungo e faticoso lavoro di mediazione possono qualificare non una parte, ma l'attività del Parlamento. Per noi la legislatura e il Governo possono andare alla conclusione naturale. È possibile; si può fare ricostruendo la collaborazione nella maggioranza e il dialogo con le opposizioni

Ma la nostra responsabilità non può significare corresponsabilità verso forzature che non condividiamo come raggiramento del *referendum*. Il Gruppo Articolo 1 non parteciperà al voto di fiducia. È la prima volta che lo facciamo; si tratta di una presa di distanza netta di cui siamo consapevoli, una scelta obbligata o l'unica possibile per non arrendersi all'accettazione in blocco o al rifiuto in blocco del decreto-legge. no, quindi, a quella che giudichiamo una forzatura sui *voucher*, contraria ai nostri valori costitutivi: la dignità del lavoro, la partecipazione democratica. Nello stesso tempo, per la responsabilità che sentiamo verso il Paese, lasciamo una porta aperta a scelte, nel metodo e nel merito, più condivise nel futuro.

l'intervento che mi ha preceduto e il fatto che non ci sia più maggioranza in questo Parlamento. C'è un Gruppo di maggioranza che ha detto che non vota la fiducia e l'ha detto con toni forti e chiari. una presa di distanza netta. Presidente, credo che lei debba informare il Presidente del Senato, perché nella prima Repubblica bastava molto meno per aprire una crisi di Governo e perché non penso che qui si abbia un Governo a tarallucci e vino per cui un giorno c'è una maggioranza e il giorno dopo

il bilancio di questi ultimi quattro anni vissuti pericolosamente dal punto di vista economico è che, almeno dal punto di vista delle riforme da fare, il Paese è rimasto al palo. Noi eravamo un Gruppo

perché esiste questo ricatto e il Governo non è libero di portare avanti le riforme necessarie al Paese e che, in un tempo lontano, avevano portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica

cento. È un encefalogramma piatto durante la gestione di Enrico Letta e leggermente migliore con il Governo Renzi, ma la prognosi resta riservata perché serve un Governo forte.

Perché non ci sono investimenti? Perché non si fa la politica per gli investimenti e si sta ad ascoltare la CGIL e la magistratura (cui si dà un potere enorme, che impedisce agli investitori stranieri di venire a investire in Italia). La malagiustizia, la malasanità la burocrazia italiana, che non si è voluto riformare in alcun modo, hanno portato questo Paese a languire. Ha tirato solo l'estero, ma in crescente affanno. Il suo contributo alla crescita complessiva è infatti diminuito dall'inizio della legislatura, passando dati spiegano l'anemia. Sulle cause relative ci siamo più volte soffermati: si tratta soprattutto delle mancate riforme *pro-growth* (orientamento alla crescita), come dicono gli economisti, a partire dalla bassa produttività aziendale e complessiva.

programmi, obiettivi e confini chiari, cosa che non esiste. Se viene meno questa spinta, la società si rattrappisce. Il piccolo cabotaggio prende il sopravvento e alimenta l'illusione che si possano separare i propri destini da quelli più generali. Eppure, qualcosa avrebbe

Nell'affondamento del Titanic non si sono salvati i passeggeri che occupavano le cabine di prima classe. Costruire un orizzonte un Governo più solidi è quindi il primo requisito. Il secondo è fare veramente i conti con l'Europa, senza levate di scudi e intemperanze, ma con la forza tranquilla che deriva dalla convinzione di essere dalla parte della ragione.

non sarà definitivamente alle nostre spalle. Ne era consapevole il Parlamento europeo quando propose alla Commissione quel periodo di sperimentazione che ora volge al termine. Ebbene, i relativi esiti sono stati negativi. Se guardiamo alla stessa dinamica del debito pubblico, possiamo constatare come esso sia cresciuto a causa soprattutto dell'austerità e non già della crisi finanziaria internazionale. Ripeto, è stata l'austerità a far crescere il debito pubblico. La spiegazione è semplice, come dimostra l'autocritica, seppur tardiva, dello stesso Fondo monetario internazione. È stato il suo capo economista, Olivier Blanchard, a dimostrare che avevamo ragione erano sbagliati, in quanto, nel predisporre le relative cure, si era trascurato di considerare l'effetto deflazionistico che l'eccesso di rigore determinava, contribuendo a deprimere oltre misura il tasso di crescita del PIL.

e vi sia più tempo per verificare sul campo i relativi risultati. Torneremmo, così, ai vincoli previsti dalla normativa in vigore, a quel margine del 3 per cento per l'indebitamento che dovremo usare in modo produttivo. E che deve usare un Governo omogeneo e forte, che abbia un programma vero e che non sia sempre sotto ricatto. Via *bonus* e prebende, ma investimenti pubblici e privati e riduzione del carico fiscale; via burocrazia, sì alla riforma della giustizia; sì, ovviamente, alla riforma di quella sanità regionale, che alimenta solo il debito pubblico. Ecco la certezza che serve per rimettere in moto il Paese; una sorta di programmazione di medio periodo che possa contare su risorse certe fin dall'inizio e non sulla benevolenza o l'elemosina, sempre un po' pelosa, di Angela Merkel o, peggio, del suo Ministro dell'economia. Propositi per il futuro: ne sono consapevole. Un Governo forte dovrà però avere la forza per cambiare pagina. Affinché questo si realizzi è però necessario sin da ora porre gli strumenti cognitivi più opportuni, contribuire a far nascere una coscienza collettiva, che è il presupposto per qualsiasi possibile riscatto, se non vogliamo che la prospettiva sia quella indicata dalle pagine, che nessuno ha letto, nemmeno i signori Ministri che siedono ai banchi del Governo, circa la diagnosi che ha fatto il Fondo monetario e di quanto scritto dal Governatore della Banca d'Italia. L'unica certezza è che l'Italia non può permettersi di crescere a quell'uno per cento che è stato indicato: sarebbe bruciare altre generazioni di giovani, alimentare una rabbia, un malcontento diffuso, sopito - come dimostrano le ultime elezioni amministrative - ma non domato. Il nostro voto sarà quindi contrario, ma non per ragioni di tattica parlamentare. Un eventuale voto favorevole suonerebbe come un avallo alle politiche anemiche fin qui seguite seguite da questo Governo debole; cloroformio distribuito a piene mani a un paziente colpito da una grave malattia. Preferiamo pertanto assumerci in pieno le nostre responsabilità, anche a costo di apparire come coloro che vanno controcorrente. Sappiamo però che almeno in questo caso il tempo è galantuomo; ci darete ragione. Ancor più importante è però che ci daranno ragione tutti coloro che non hanno bisogno di analisi sofisticate per capire la reale natura di questa crisi, che è ancora lungi dall'essere superata, perché la vivono quotidianamente, sulla propria pelle e su quella delle proprie famiglie, gli italiani che vogliono le riforme della sanità, della giustizia, la sburocratizzazione soprattutto per permettere gli investimenti stranieri in Italia. Altrimenti noi saremo costretti a perire. [MAURO

Una manovra che è andata ad affondare a piene mani nell'individuazione di tre nuove tasse e capitoli da cui attingere risorse. Dal punto di vista della redistribuzione, abbiamo invece assistito all'ormai solita, per questa maggioranza a traino del

ci saremmo attesi - anche per compiacerci eventualmente della volontà del partito di maggioranza di questo Parlamento

dello sviluppo. Si è detto in altra sede e altra occasione che uno degli elementi fondamentali dello sviluppo sarebbe dovuto essere il Mezzogiorno d'Italia. Si è detto, anche da colleghi intervenuti prima di me, che potrebbe esservi una manovra più complessiva, con un prossimo decreto sul Mezzogiorno che individui le ZES, le zone economiche speciali, speciali, e gli strumenti di una fiscalità di vantaggio. Ebbene, come fa un Governo a non avere una visione complessiva, globale e unitaria di un problema? Se si crede veramente che lo sviluppo dell'intero Paese passi soprattutto e fortemente attraverso lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, come si fa da un lato a individuare strumenti come le zone economiche speciali e, dall'altro, a sottoscrivere i patti delle nuove vie della seta, individuando l'asse dello sviluppo per questa per questa vie nei porti di Livorno e Trieste? Infatti, così facendo, si sposta completamente il baricentro dei commerci con i nuovi colossi della produzione mondiale, che sono l'India e la Cina, totalmente al di sopra dell'asse del Mezzogiorno d'Italia, con ciò non assolvendo nemmeno a quella normalissima logica di trarre il maggiore profitto possibile da questi commerci. Le nuove vie della seta attraversano il Mediterraneo in virtù del Canale di Suez, che ha dovuto raddoppiare la possibilità di passaggio delle navi proprio per l'aumento delle produzioni. Ebbene, anziché individuare i porti del Sud, anziché individuare la Sicilia come naturale piattaforma logistica naturale del Mediterraneo, costringeremo le grandi navi che provengono dal Sud-Est asiatico, dalla Cina e dall'India a entrare nell'Adriatico e nel Tirreno e poi ritornare nel Mediterraneo, perché con navi più piccole possano rifornire le altre zone del commercio europeo e africano. Con ciò il Governo dimostra chiaramente di non avere minimamente a cuore lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Con ciò il Governo dimostra di aderire più alle logiche di tipo imprenditoriale e finanziario che a quelle dello sviluppo complessivo. Potremo creare tutte le zone economiche speciali che vorremo, ma se non ci saranno i motivi per la produzione e le occasioni

una propria presenza, continua a pagare per scelte di un Governo nazionale assolutamente lontano e nemico rispetto alle esigenze di questo territorio, anche per altri aspetti che riguardano

che pure è stata promessa più volte. Ma di cosa pensate debba vivere il nostro Paese? Se la logistica e i commerci devono essere tagliati fuori, se la nostra agricoltura, anche quella di avanguardia, non può trovare protagonismo per via della concorrenza sleale, come pensate di poter di poter salvare o contribuire a far rinascere questo Mezzogiorno d'Italia? Voi siete senza un progetto. In questi anni di governo avete seguito soltanto l'alta finanza e ne sono prova gli episodi di queste ultime settimane, perché il vostro problema sono state sempre le banche; non le banche come strumento per lo sviluppo, ma come alta finanza che deve compensare se stessa e deve sopravvivere. Ma non vi rendete conto che di banche dovremmo parlare per quanto riguarda i problemi dell'accesso al credito, anziché

Ritroviamo nella soluzione dell'ILVA lo stesso gruppo Marcegaglia che troviamo invischiato nei debiti del Monte dei Paschi di Siena e lo ritroviamo in una posizione di apparente partecipazione dell'industria italiana al salvataggio di un polo industriale come quello dell'ILVA di Taranto, pronto a sfilarsi a vantaggio del sistema bancario e finanziario. Di finanza non si vive; di finanza si arricchiscono soltanto pochissime persone. È il lavoro che salva il nostro Paese! È la produzione che salva il nostro Paese! E lavoro e produzione e reddito in Italia lo fanno le piccole e medie imprese e le famiglie; piccole e medie imprese e famiglie che sono assenti da questo decreto-legge che voi chiamate manovrina e che definite come strumenti per agevolare lo sviluppo del Paese. Paese. Le nuove tasse che introducete non vanno nella direzione del sostegno a questi settori, che sono fondamentali; non vanno al sostegno dell'agricoltura. Mentre noi parliamo, provvedimenti di grande semplicità potrebbero aiutare, alleviare lo sconforto e la mancanza assoluta di fiducia che sta colpendo la nostra piccola e media impresa. Cito, ad esempio, la questione delle aste giudiziarie per le case. Vengono tolte le case ad uso abitativo per 17-20.000 euro a persone che non hanno potuto pagare, in un momento di contingenza economica sfavorevole, i debiti con le banche. E mentre le banche possono cedere i loro crediti cosiddetti deteriorati al 7, 8, 9 per cento, ai poveri disgraziati che incappano nelle procedure bancarie non solo chiediamo tutto il ristoro, ma mettiamo anche all'asta le loro case con tutte le spese di procedura. Su questi temi non possiamo abbassare assolutamente la guardia. Nel dire a questa Governo e a questa maggioranza che hanno abbandonato la strada dei bisogni reali del Paese,

negando la fiducia su questo provvedimento, rimarchiamo che il nostro Paese ha bisogno di un programma produttivo che consideri l'Italia tutt'una, da Trieste fino a Capo Passero, che abbia la consapevolezza che senza

Vice Ministro, colleghe e colleghi, la manovra correttiva è coerente con le politiche di risanamento dei conti pubblici e con l'obiettivo di intervenire sui limiti strutturali che hanno determinato una tendenza di lungo periodo certamente segnata da una crescita debole e intermittente. È stato comunque importante che la correzione dei conti pubblici di 3,4 miliardi, pari allo 0,2 per cento del PIL, sia avvenuta rispettando l'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale. È fondamentale che ciò sia avvenuto mantenendo l'impegno a non intervenire con aumenti dell'IVA o con l'incremento delle accise sui carburanti nel 2018 a copertura della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Il consolidamento dei risultati ottenuti per quel che riguarda il debito e la contrazione del *deficit* pubblico sono orientati alla crescita, in primo luogo, con una riduzione del carico fiscale, con il sostegno agli investimenti e con altre misure strutturali. Condividiamo la strategia che prevede il dimezzamento dell'aggiustamento strutturale per il 2018 pari allo 0,3 per cento del PIL e, grazie a una migliore crescita del prodotto lordo, ciò consentirà di prevedere che la prossima legge di bilancio sarà una manovra equa, in grado di garantire l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, senza che vi sia un'inversione di tendenza delle misure di risanamento, e contestualmente potrà aprire opportunità di bilancio in grado di sostenere i redditi, di finanziare più ampi e maggiori elementi di *welfare* e, fattore decisivo, di intervenire sul costo del lavoro (il cosiddetto cuneo fiscale) per incrementare la produttività e la competitività del mondo produttivo italiano. Le incisive politiche di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale hanno prodotto risultati significativi e liberato risorse a favore di politiche industriali e sostegno ai redditi e alle imprese, mentre non è affatto irrilevante che complessivamente la pressione fiscale sia scesa

Si confermano con la manovra le linee e i dati guida indicati dal Governo nel Documento di economia e finanza per il 2017. Parimenti, condividiamo la decisione di stimolare investimenti selettivi in settori di produzione coerenti con la strategia Industria 4.0 attraverso ulteriori agevolazioni fiscali. Nel DEF il Governo ricordava come la riduzione di imposte sia avvenuta in modo strutturale con la revisione delle componenti della base imponibile di alcune imposte, in particolare IRAP (per il e IMU (su macchinari e impianti imbullonati) nel 2016, e la riduzione delle aliquote IRES nel 2017. Riteniamo fondamentale l'obiettivo di sostenere la crescita mediante il completamento e il rafforzamento delle riforme. È molto importante insistere, con riferimento a Industria 4.0, su una politica industriale che abbia al centro il rinnovamento tecnologico, lo stimolo della competitività del sistema impresa e l'esigenza di continuare sulla strada delle privatizzazioni attraverso un *iter* equilibrato e con misure strutturali in una prospettiva di medio termine (equilibrio nelle scelte e negli obiettivi di finanza pubblica, dunque). Si consolida una direzione di marcia verso il risanamento di conti con il *deficit* in contrazione costante tra il 2014 e il 2016, ma con una velocità di marcia adeguata alla necessità di sostenere la ripresa dell'economia reale. È in quest'ambito che riteniamo fondamentale intervenire sia sul piano fiscale sia su quello economico, a sostegno delle politiche sociali per la famiglia. Rilevante in questa manovra correttiva è peraltro l'insieme di misure previste a favore degli enti territoriali, a cui vengono assegnate nel periodo 2016-2020 risorse aggiuntive per oltre 2 miliardi, uno dei quali viene assegnato già nel 2017. di un'inversione di tendenza rispetto agli anni nei quali gli enti locali hanno dovuto amministrare sulla base di minori risorse in ragione dei vincoli di finanza pubblica. In campo fiscale sono apprezzabili diverse misure, tra le quali figurano l'istituzione di una *web tax* transitoria sui colossi di Internet; la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa; d'impresa; la modifica della disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale; la modifica della disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi d'incremento dell'efficienza energetica nei condomini; e il contrasto all'evasione fiscale. Riteniamo sia stato compiuto un grande passo a favore dell'emersione spontanea delle basi imponibili e per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti,

Come Gruppo per le Autonomie esprimiamo soddisfazione anche per la disposizione che prevede l'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano dai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Colgo l'occasione per ringraziare il Governo per aver accolto diversi ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo e in particolare quello che estende le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione e quello sull'Università di Trento. Ci auguriamo che la prossima legge di bilancio contenga le misure *ad hoc* per quest'agevolazione e traduca in disposizioni anche gli altri impegni assunti.

Le disposizioni introdotte nel decreto-legge sul tema migliorano la situazione, sia in ordine alla esigenza di evitare possibili abusi o violazioni, sia in relazione a fattispecie che richiedono forme di lavoro di particolare flessibilità: si delinea finalmente - così come alcuni tecnici lo hanno classificato - un contratto di lavoro che stabilisce minimi retributivi orari, molto diversi quindi dai *voucher* abrogati e, per la prima volta, si introduce una forma di salario minimo. Il contratto di prestazione occasionale rappresenta per le microimprese, fino a cinque dipendenti, uno strumento sicuramente adeguato e semplificato. Analoghe considerazioni debbono valere per l'introduzione del libretto telematico prefinanziato a disposizione delle famiglie in ordine agli asili nido, al *baby sitting* e alla retribuzione di attività di assistenza o a quelle, senza fini di lucro, gestite dai privati. In conclusione, i dati economici confermano che non vi è dubbio che occorra operare strutturalmente per compiere progressi oltre la crescita moderata e ancora non sufficiente, soprattutto se confrontata con le altre dinamiche europee. Condividiamo però che vi siano ulteriori margini di miglioramento nelle misure di riqualificazione della spesa. Riteniamo che il tema fiscale abbia costituito e sia il punto discriminante ai fini della crescita e che tale obiettivo debba essere compatibile con una prospettiva discendente del rapporto tra debito e PIL. Dobbiamo sempre ricordare, infatti, che abbiamo un enorme debito pubblico. Ebbene, a gennaio le stime di crescita erano dello 0,7 per cento. Oggi le previsioni di crescita

ma mettono in evidenza come il lavoro svolto fino ad oggi e che dovrà necessariamente e con forza continuare in futuro paghi, ad iniziare - così ci auguriamo - dalla prossima legge di bilancio, che certamente dovrà essere equilibrata e siamo certi che non solo consoliderà i conti pubblici, ma continuerà a incentivare il cammino della crescita economica. Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie - Partito socialista italiano voterà convintamente la fiducia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in premessa è bene parlare dello scopo e dell'obiettivo principale del decreto-legge in esame: esso nasce per una correzione sui conti pubblici richiesta dall'Unione europea, per portarci agli obiettivi di medio termine, dai quali si registra per il nostro Paese uno scostamento di poco meno dello 0,2 per cento. Infatti, la correzione sull'indebitamento netto che si realizza nella manovra è di 3,1 miliardi di euro. di un risultato importante, che raggiungiamo senza aumentare la pressione fiscale e senza fare tagli draconiani alle spese per i servizi ai cittadini. Com'è noto, la maggior parte della copertura di tale decreto arriva dall'estensione della platea dello *split payment*, misura molto criticata in passato. Riprendendo il dibattito svolto l'anno scorso

è stata importante e l'ampliamento porterà ulteriore emersione. Inoltre, abbiamo approvato tagli alle spese improduttive dei Ministeri e una tassazione aggiuntiva sul sistema del gioco. Queste sono le voci fondamentali da cui si reperiscono le risorse non solo per raggiungere quella correzione sui conti pubblici di cui ho parlato, ma anche per realizzare altre misure molto importanti. Voglio ricordare che, solo per l'annualità 2017, con la manovra, rifinanziamo le spese per il terremoto nel Centro Italia di circa 700 milioni di euro. Oltre a tale fondamentale aggiunta di risorse, un'altra norma che implementiamo, grazie anche al lavoro della Camera dei deputati, prevede l'aumento complessivo della dotazione finanziaria in capo alle Province di quasi 400 milioni di euro, rispondendo a una questione posta al Parlamento negli ultimi mesi dai rappresentanti delle istituzioni territoriali di tutti i colori politici. In questo contesto riusciamo a realizzare, oltre alla correzione dei conti, anche i primi passi del percorso di neutralizzazione parziale delle clausole di salvaguardia per il 2018 e 2019. È chiaro che rimane un grandissimo sforzo da fare: devono essere ancora neutralizzate clausole per circa 15 miliardi per scongiurare l'aumento delle tasse e, in particolare, l'aumento dell'IVA, che sarebbe disastroso in questo momento per il Paese. È uno sforzo che dobbiamo sostenere, naturalmente in un negoziato che deve continuare con l'Europa e deve essere costante. Come Gruppo Alternativa Popolare, rivendichiamo il continuo dialogo costruttivo nelle sedi europee come uno dei maggiori risultati di questo Gruppo, purtroppo non riconosciuti né - da una parte - da chi ci dice che dovremmo essere più rigorosi con l'Europa, né - dall'altra - da chi ci dice che dovremmo uscire dall'Europa. Crediamo che la correzione che oggi facciamo sui conti pubblici, proprio per rispettare gli obiettivi di medio termine e continuare in una strada di serietà, di rispetto in ordine alle regole europee, ci metta nella condizione politica di sedere al tavolo dei negoziati in una posizione di ancora maggiore credibilità per avere dei risultati simili, se non migliori, di quelli che abbiamo già ottenuto negli anni passati. Sono risultati - lo ricordo - che ci hanno consentito di approvare misure innovative e fondamentali per il rilancio e la crescita economica, come gli sgravi contributivi, l'abolizione dell'IRAP sul lavoro, il superammortamento delle misure per il Piano Nazionale Industria 4.0. Sono tutti strumenti varati proprio grazie a una flessibilità che questo Governo ha ottenuto dall'Europa. Ebbene, io credo che dobbiamo continuare su quella strada, perché oggi, grazie anche a questa correzione, abbiamo tutta la legittimità per chiedere ancora dei margini di flessibilità di bilancio anche per il 2018. Dobbiamo sfruttare appieno tutte le possibilità che i trattati contengono per capitalizzare le nuove positive tendenze del sistema economico italiano certificate dall'ISTAT e, in tal senso, si è registrata un'importante apertura parte di autorevoli autorità europee. Da questo punto di vista, è imprescindibile che ci sia un Governo a trattare e a negoziare su questi temi, e sia in grado di presentare una legge di bilancio e di affrontare una sessione di bilancio seria. Noi abbiamo avuto un aumento dell'occupazione, negli anni in cui abbiamo governato, di circa 850.000 unità. Abbiamo un aumento del PIL che è maggiore di quello stimato. È un percorso molto lento di miglioramento, ma - ripeto - i dati ci dicono che è la strada che dobbiamo seguire. Per questo ritengo e ribadisco assolutamente irresponsabile pensare a scenari politici destabilizzanti, proprio nel periodo della gestione della manovra, sia in Italia che in Europa. Mi soffermo ancora, signor Presidente, su due aspetti che sono stati oggetto del lavoro del Parlamento. Il primo, già venuto in rilievo in più sedi, è quello della questione dei *voucher*. Noi abbiamo votato l'ipotesi proposta dal Governo sulla reintroduzione parziale di un contratto per la gestione del lavoro occasionale. però, che quella misura sia assolutamente deludente, insoddisfacente e non copra tutte le esigenze del tessuto produttivo e imprenditoriale. L'abbiamo votata perché comunque è un passo in una direzione per noi condivisibile: è una misura che va a coprire almeno alcune delle esigenze che abbiamo lasciato scoperte con il decreto di abolizione dei *voucher*. I *voucher* hanno avuto un grande utilizzo. Quando vediamo che una misura ha una grande risposta, per noi è un successo, e non uno strumento da eliminare. Pur rimanendo una piccolissima percentuale all'interno dell'intero monte ore lavorate nel nostro Paese, quale fenomeno assolutamente marginale, rispondeva a esigenze importanti. Per sintetizzare, siamo assolutamente contrari all'approccio culturale del limite di personale a tempo indeterminato dentro le aziende. Il lavoro occasionale

Questo è discriminante, divide il mondo delle aziende, mette un paletto che può essere un problematico balzello: è chiaro che un'azienda avrà problemi ad assumere la sesta la sesta persona e naturalmente avrà convenienza a rimanere con cinque dipendenti. Quindi, da questo punto di vista, pur considerando estremamente deludente quel risultato, abbiamo votato perché pensiamo che sia comunque un piccolo passo avanti. Per chiudere, Presidente, vorrei dedicare poche riflessioni alla questione del terremoto e del sisma nell'Italia Centrale. Nel decreto-legge sono ricomprese due misure importanti: una è rappresentata dal rifinanziamento per 700 milioni sul 2017 (e un miliardo a regime)

Noi abbiamo apportato due modifiche importanti all'impianto del decreto-legge. La prima prevede l'aumento del finanziamento e la copertura per il cosiddetto danno indiretto, sostanzialmente raddoppiata. Si tratta di una possibilità che risponde alle esigenze manifestate fortemente dalle aziende, soprattutto in particolari settori, che erano state molto penalizzate. La seconda fa riferimento alla possibilità, a *budget* fermo, di finanziare anche le ricostruzioni complete di edifici e quindi, la possibilità di ristrutturare abbattendo e ricostruendo gli edifici completamente, contribuendo in modo sostanziale alla maggiore qualità del nuovo patrimonio edilizio. Il decreto-legge al nostro esame provvede ad affrontare situazioni diverse riconducibili alla necessità e urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; a introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; inoltre - come detto - il provvedimento è diretto a intervenire per introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 contiene una sintesi di misure di risanamento dei conti pubblici e di interventi per rilanciare la crescita e gli investimenti che costituiscono le basi fondamentali per lo sviluppo del sistema Paese. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole di fiducia al Governo sul decreto-legge da parte del Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa.

A novembre del 2016 la Commissione dell'Unione europea ha chiesto di assumere misure aggiuntive per il 2017, e cioè di prevedere una correzione, entro il mese di maggio, del disavanzo strutturale di bilancio previsto per il 2017, di almeno lo 0,2 per cento del PIL, pari a circa 3,4 miliardi di euro. Per chi sa leggere i numeri, ciò significava una sanzione relativa alle scelte operate da Renzi nella legge di bilancio 2017, costruita per rispondere anche alle promesse elettorali per il *referendum* del 4 dicembre, sonoramente bocciato dagli elettori italiani. delle tensioni e delle contraddizioni di questa maggioranza, ostaggio di veti incrociati in perenne campagna elettorale, il Governo, ancora una volta, ha scelto la decretazione d'urgenza, impedendo al Parlamento di esercitare pienamente le sue prerogative istituzionali. E così ci troviamo di fronte non ad una manovrina ma ad una sorta di mostro giuridico del tutto eterogeneo, con buona pace delle promesse di semplificazione della ministra Madia e dell'ex *premier* Renzi: 465 sobrie pagine in cui siete riusciti ad infilare di tutto, tranne misure efficaci per uscire dalla crisi. Siamo 7 o 8 punti sotto il PIL del 2007; la disoccupazione è ancora sopra l'11 per cento e il CENSIS, proprio in questi giorni, ha confermato che più di 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per mancanza di soldi, e ci sono ancora quattro milioni e seicentomila persone povere che vivono in miseria. Dopo aver annunciato, con l'ormai famoso *tweet*, che si mandavano a casa 3.000 politici delle Province, asserita fonte di tutti gli sprechi, per chiuderle ecco arrivare risorse per le Province e Città metropolitane per garantire lo stipendio ai dipendenti, l'edilizia scolastica (ma, a proposito, non doveva passare tutto alle Regioni?), la manutenzione delle come si fa? Si dà la possibilità di fare cassa con gli *autovelox* e utilizzare quei soldi per la viabilità e polizia locale in deroga alla legislazione vigente, che impone di devolvere una quota non inferiore a un quarto dei proventi alla sicurezza stradale (segnaletica e cartellonistica). E, in virtù di questo, le amministrazioni potranno destinare i proventi delle relative multe per la copertura di costi di bilancio piuttosto che per incrementare la sicurezza sulle strade. Eppure, io ricordo ancora un ex Presidente della Provincia di Firenze che si indignava fortemente contro i Comuni che mettevano *autovelox* non segnalati solo per fare cassa. In questa manovrina, sono tanti gli interventi *ad personam.* All'articolo 62 si inserisce un provvedimento che è arrivato con singolare tempismo proprio quando era in corso la conferenza dei servizi per la costruzione dello stadio di Tor di Valle. Si dà la possibilità infatti ad un organismo tecnico, che decide a maggioranza, di approvare una variante al piano regolatore, in barba alla competenza del consiglio comunale e si introduce la possibilità di edilizia residenziale nella costruzione degli impianti sportivi, e non solo degli stadi. Ricordo che a inizio legislatura alcuni parlamentari hanno decantato la norma

residenziale, persino utilizzando l'immagine di Totti per convincere la politica. Ma - ahinoi - abbiamo visto che l'immagine di Totti è più che sfruttata da molti politici.

parlando di persone che sanno già che presumibilmente quel contenzioso lo perderanno; sono stati già giudicati di fatto evasori in primo grado e adesso, con un colpo di spugna, pagando solo ed esclusivamente quanto dovuto, senza penali, senza aggravanti e ulteriori gravami, tornano puliti pur con una condanna in primo grado. In questi anni abbiamo discusso molto di una legge su AFAM e statizzazione degli istituti pareggiati. Improvvisamente si cambia rotta

tutele per il personale, tutele per i precari degli statizzati e i precari dei licei musicali e le accademie. E naturalmente i Comuni, quegli enti locali che in questi anni hanno visto abbattersi con ferocia la scure dei tagli anche nella cultura, dovranno farsi carico dei debiti pregressi degli istituti da statizzare. Devo dire che non si sa se ridere o piangere. E cosa accade agli istituti i cui Comuni non potranno farsi carico dei debiti? Ma si sa: la campagna elettorale è vicina ed è meglio un miraggio per continuare a garantire almeno le risorse necessarie, pena la chiusura; per il resto si vedrà, tanto nel frattempo alcuni conservatori iniziano a chiudere e agli investimenti economici e culturali per far sopravvivere e crescere istituti dove si continua a produrre musica e arte, grazie al sacrificio e all'abnegazione di decine di musicisti e di artisti, ci penserà qualcun altro. Ovviamente, non poteva mancare la sanatoria per i direttori dei musei. Eppure, il TAR vi ha ricordato che le leggi vanno rispettate, e non solo quelle approvate con la fiducia in fretta e furia con ansia di prestazione degna di miglior causa, ma anche quelle di cui avete persino perso traccia. poi abbiamo gli otto milioni al teatro Eliseo, emendamento che era stato ritirato dal mille proroghe. A quale criterio oggi corrisponde un finanziamento fuori FUS, proprio mentre in queste ore si discute in Commissione la legge sullo spettacolo dal vivo e senza un serio intervento economico e finanziario sull'intero sistema teatrale che da anni deve fare i conti con la riduzione di risorse. Si aiuta un teatro privato in difficoltà? Bene, allora sarà un principio e un precedente inderogabile da utilizzare per tutte le realtà del mondo dello spettacolo che hanno i bilanci in rosso, soprattutto per quelli pubblici, dove troppo spesso si licenziano i lavoratori per far quadrare i bilanci e poco i *manager.* mancano ancora i soldi per ristrutturare il teatro Valle, il più antico teatro di Roma, di proprietà totalmente pubblica, che conta solo un quarto delle risorse necessarie. Noi non saremo in silenzio dinanzi alla violazione dell'articolo 9 della Costituzione. Infine, questa manovra lascerà il segno sopratutto per la grave scelta di reintrodurre i *voucher:* un'operazione grave, furba, a dir poco anticostituzionale, Voi oggi reintroducete i *voucher* tagliati in fretta e furia a marzo per non passare dal vaglio di un *referendum* per il quale la CGIL aveva raccolto oltre 3 milioni di firme; un voto che si sarebbe dovuto svolgere a pochi giorni dalle elezioni amministrative era troppo pericoloso. Votare o dare assenso a questa manovra anche solo uscendo dall'Assemblea vuol dire mettere in discussione i principi costituzionali. Siamo dinanzi a un arrogante esercizio del potere. Ma come si pensa di recuperare la fiducia dei cittadini nei

si inventa un decreto-legge per non far votare i cittadini, decreto-legge che abbiamo votato anche noi dell'opposizione, e poi alla prima occasione si reintroducono i *voucher* in maniera a dir poco subdola, invocando anche che si tratti di altro? un vero furto di democrazia e di un grave precedente anticostituzionale: il tutto in nome dell'emersione del lavoro nero, tralasciando di dire, in modo doloso, che esistono forme contrattuali variegate, che sempre voi avete votato, per i lavori stagionali o intermittenti e non è necessario sostituire contratti già precari con altri ancora più vergognosi. Aggiungo che la vostra operazione è particolarmente grave perché, con le vostre leggi, state modificando la cultura I giovani sono ormai rassegnati alla precarietà, assuefatti e incapaci di reagire, al punto che diventa normale accettare di essere pagati dietro presentazione di scontrini; rassegnati a un futuro senza lavoro e questo è un danno per tutta Siamo quindi dinanzi a un attacco gravissimo al nostro sistema democratico ma in perfetta sintonia con le vostre presunte riforme di questa legislatura, caratterizzate tutte dal tono autoritario. Dalla legge Delrio sulle Province, alla riforma costituzionale, passando per il *jobs act* e la legge buona scuola, nonché la vostra bozza di legge elettorale, l'obiettivo manifesto e non più nascosto è l'azzeramento degli spazi e della partecipazione democratica in nome dell'ideologia dell'uomo forte o della donna forte sola al comando. Noi di Sinistra Italiana voteremo voteremo contro questo decreto-legge in modo chiaro e coerente e sabato 17 giugno saremo in piazza con la CGIL, a ricordarvi che la democrazia è intoccabile.

l'eccesso di *deficit* pubblico attualmente esistente; una correzione strutturale di almeno lo 0,2 per cento del PIL (circa 3,5 miliardi) che non permette al nostro Paese di rimanere in linea con il percorso di convergenza verso il pareggio di bilancio previsto dai trattati europei. Stiamo, dunque, parlando di una manovra correttiva dei conti pubblici chiesta da Bruxelles, che avrà un impatto recessivo inevitabile. Si giustifica il decreto-legge in esame affermando che questo intervento si muove in uno spazio stretto, tra le esigenze di consolidamento fiscale e di sostegno alla crescita. Perché invece non ammettete che le ragioni per cui l'Italia non prospera e non cresce veramente - in termini soprattutto sociali - stanno anche e soprattutto nelle scelte europee? Perché non confessate il vero peccato originale, ovvero che l'Europa - imponendo una dose massiccia di austerità nella forma di tagli alla spesa pubblica - ha fallito miseramente, riuscendo a far aumentare le diseguaglianze, la povertà assoluta e aumentando la divergenza? Né l'austerità né le riforme strutturali vere o presunte fino ad oggi sono riuscite a riportare quella prosperità nel nostro Paese e ciò che è peggio è che aggravano la recessione. Ma, soprattutto, l'errore principale che è stato e si continua a compiere è focalizzare tutta l'attenzione sui disavanzi di bilancio, tanto da formulare una diagnosi sbagliata del problema. La cura che ci state propinando è sbagliata, è devastante e fallimentare. A poco serve dire che queste politiche in futuro faranno stare meglio tutti o devono essere accettate dai cittadini, i quali - a vostro modo di dire vedranno i vantaggi e non subiranno solo conseguenze negative. Non è così, non è vero. La vera vostra preoccupazione è riuscire a mettere in campo azioni per evitare ricadute negative sull'Unione economica e monetaria. L'Italia continua a presentare squilibri macroeconomici eccessivi, a partire dalla dinamica ancora debole della produzione, dall'elevato volume di crediti deteriorati e dalla forte disoccupazione. Inoltre, le manovre recessive imposte per soddisfare Bruxelles hanno prodotto l'effetto opposto, cioè l'aumento del il rapporto debito/PIL. Ciò che stride di più è che questo Governo nonostante tutto abbia deciso di proseguire con la logica delle manovre, ovvero con quella serie di operazioni necessarie per il funzionamento della macchina economica di un Paese che è arrivato al collasso, nonostante qualcuno faccia ancora credere che stia crescendo in termini di PIL. Stiamo parlando, quindi, di una manovra per correggere i conti che voi avete sbagliato e che l'Europa ci chiede di sistemare. Eppure, non credo che l'Europa abbia chiesto di sistemare i conti inserendo - ad esempio - il comma 4 all'articolo 22

presso pubbliche amministrazioni, che prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e l'attribuzione di gettoni di presenza fino ad un massimo di 30 euro a seduta. In sostanza, avete pensato bene di stabilire che non rientrano tra i suddetti incarichi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte di pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Non posso, poi, non rimarcare alcuni punti di questo provvedimento. Intanto rimangono confermate le clausole di salvaguardia fiscali che avete fissato, seppure in parte ridotta, al 1° gennaio 2018, per un importo più contenuto di 15,2 miliardi anziché 19,6. Sul punto se ne riparlerà a ottobre. Vediamo se l'impegno assunto riuscirete a onorare veramente. Noi abbiamo più di un ragionevole motivo per pensare che non ci riuscirete se non con qualche altro taglio, ma purtroppo sempre a scapito dei cittadini che non lo meritano. Quanto alla collaborazione volontaria, vorrei ricordare che vi hanno aderito davvero in pochi. Pertanto, sarà difficile raggiungere gli introiti da voi previsti, a maggior ragione visto che le vostre previsioni non solo sono improbabili, ma soprattutto non sono certe.

I 600 milioni previsti nella manovra per il salvataggio di Alitalia vengono chiamati prestito ponte o finanziamento. Il motivo di questa elargizione si fonda sulla volontà di salvare l'occupazione del personale della *ex* compagnia di bandiera. Almeno questo è il motivo di facciata. Quello vero, invece, si sostanzia nella necessità di dovere coprire i buchi e le perdite causati dalla politica a un'azienda che doveva essere il nostro fiore all'occhiello. Dietro a questa scelta purtroppo manca un valido e fattibile piano industriale, ma si sa: siete soliti fare tutto senza considerare le cause, le conseguenze, ma soprattutto gli impatti in termini economici. Tanto, a chi importa se poi a Bruxelles vengono aperte procedure di infrazione per aiuti di Stato illegittimi? L'importante non sono le infrazioni, ma poter sbandierare a tutti che la questione Alitalia è stata da mesi al centro dei tavoli tecnici dei vostri Ministeri. Non vi inutile nascondere il nostro rammarico nel veder ridurre i fondi sul trasporto pubblico locale per un ammontare pari a 135 milioni di euro, nel mentre avete pensato bene di prevederne 97 a garanzia della Ryder Cup. A fronte di tutte queste scelte del Governo, viene da chiedersi: ma dove sono andate a finire quelle politiche che garantiscono la prosperità, intesa non semplicemente come incremento del PIL, ma come una prosperità condivisa, come una prosperità condivisa, in cui i valori democratici vengono onorati e rispettati e si promuovono la solidarietà e la coesione sociale? Avete affermato più volte che coniugare correzione dei conti pubblici a misure di sviluppo e sostegno dell'economia è abbastanza complicato. Questo è certo; ma, dato che gli errori compiuti in questa legislatura dall'Esecutivo sono innumerevoli e riguardano molteplici aspetti della vita di noi cittadini, forse è giunto il momento di fare un'analisi più approfondita e ampia prima di commetterne altri, magari valorizzando veramente il dibattito parlamentare. Dato che siamo certi che per il futuro farete fatica a evitare altri sbagli, io e il Gruppo politico cui appartengo esprimiamo un no convinto al voto di fiducia richiesto da questo Governo.

il decreto-legge in discussione, giunto blindato dopo le tante modifiche apportate dalla Camera dei deputati, mortifica questo ramo del Parlamento, costringendolo a non poter affrontare un esame compiuto e a dover prendere atto che ci si trova di fronte a un testo non emendabile. Nonostante le nostre proteste, al Senato viene nuovamente impedito di entrare nel merito del testo, così come già accaduto negli scorsi mesi sulla legge di bilancio e sul cosiddetto decreto fiscale. Andiamo avanti a colpi di fiducia e il nostro ramo del Parlamento vede costantemente sminuito il proprio ruolo. Il dibattito ci consente però di lasciare agli atti un'analisi sia del testo, che degli errori di politica economica replicati, anche ora, da questo Governo, sulla medesima scia del Governo precedente.

La sterilizzazione è temporanea, rinviando solamente l'aumento al 13 per cento al 2020. In termini di copertura finanziaria, quest'operazione vale 3,5 miliardi di euro. Si tratta di un intervento dopo il quale rimangono comunque in piedi più di 73 miliardi di clausole fiscali

Questo è lo stato dei fatti, in attesa che gli annunci superino ovviamente gli atti parlamentari. Questi elementi sono in grado di ridurre la fiducia dei consumatori e deprimere i consumi, venendo meno il potere d'acquisto della gente, che potrebbe quindi essere generato solo e soltanto da un'importante riduzione delle imposte sui redditi. La valutazione sui quattro anni di Governo di centrosinistra - dal 2014 al 2017 - può quindi essere fatta serenamente, numeri alla mano. delle imposte sui redditi. La valutazione sui quattro anni di Governo di centrosinistra - dal 2014 al 2017 - può quindi essere fatta serenamente, numeri alla mano. La diminuzione delle tasse, fatta soprattutto con i vari *bonus,* vale 49 miliardi di euro, mentre l'aumento delle tasse vale 57 miliardi di euro. Quindi, vi sono 8 miliardi di maggiori imposte a carico dei cittadini italiani, e non per effetto di automatismi connessi alla crescita, seppur modesta, del PIL, ma legati a scelte di politica economica. Al contrario, continua a mancare una seria revisione della spesa pubblica, che in questa manovrina vede tagli per meno di 300 milioni di euro. Siamo così a un totale di circa 44 miliardi di euro di riduzione di spesa in quattro anni, cui sono però corrisposti aumenti della spesa per circa il doppio. E come si finanzia questa differenza? Si finanzia attraverso il ricorso all'indebitamento netto, che rimane oltre i 35 miliardi nel 2017, anche se con questa manovrina viene ridotto di 3,5 miliardi. Siamo Siamo in presenza di una politica di correzione dei conti pubblici che contiene interventi ancora ipercentralisti, dove continuano a giocare il ruolo della cenerentola tutti i livelli di governo del territorio. Le misure qui introdotte sono volte a creare nuovi spazi finanziari o ampliare risorse, dopo essere arrivati all'impossibilità di garantire servizi essenziali ai cittadini. Ci riferiamo alle funzioni fondamentali degli enti di area vasta, quali quella di provvedere ai circa 130.000 chilometri di strade o ai 5.100 edifici scolastici o dare assistenza ai 234.000 alunni disabili. Ora, attraverso una restituzione temporanea di 180 milioni di euro per il 2017 e il 2018, si sta cercando di rattoppare una riforma pasticciata delle Province - presenti in Costituzione, ma non nella cosiddetta legge Delrio - dopo i tagli di 5 miliardi e duecento milioni degli ultimi tre anni. per cento della manovrina si basa, quindi, sulla crescita delle tasse. L'incremento delle imposte rappresenta sicuramente un aumento della pressione sul sistema produttivo, sia sulle imprese, che sui liberi professionisti. Sono infatti davvero poche le iniziative in loro favore in questa manovrina, che non compensano certamente l'incremento del carico fiscale qui previsto. E proprio il provvedimento in esame, resosi necessario per correggere di 0,2 punti percentuali il rapporto *deficit*-PIL, dal 2,3 al 2,1, lo fa aumentando le entrate per un importo di 2 miliardi e 800 milioni e riducendo la spesa per 300 milioni. La regola è certa: finché c'è *deficit*, il debito sale. Ed infatti il debito italiano continua a salire. Proprio qualche minuto fa, un'agenzia di Banca d'Italia lo stima a 2.270 miliardi. È aumentato di 10 miliardi rispetto al mese scorso, con un rapporto debito-PIL questa manovra viene leggermente corretto il livello massimo del saldo netto da finanziare. Così come viene corretto il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ridotto di 2 miliardi e 415 milioni, rispetto all'incremento di 20 miliardi preventivato dal decreto cosiddetto salva banche. Va detto che comunque cresce di 17 miliardi e 585 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017. Manca ancora un sostegno importante e strutturale agli investimenti, necessario a far crescere l'economia, a creare posti di lavoro stabili e a produrre un clima di fiducia nella gente, che - permettetemi il linguaggio informale - li induca a togliere da sotto il mattone. È necessario quindi continuare a sostenere il risparmio della gente, ove indirizzato a investimenti nell'economia italiana, fatta da piccole e medie imprese, che hanno un rapporto ancora molto critico con l'accesso ai finanziamenti bancari, come hanno iniziato a fare i PIR. La formula zero tasse a chi investe per più di cinque anni sostenendo le Mid Cap italiane funziona. Risulta quindi appropriata la norma che estende questa forma di investimento anche alle casse di previdenza e ai fondi pensione. Per questa particolare eccezione c'è stato un grande apporto di Forza Italia alla Camera dei deputati. Siamo purtroppo ancora molto indietro sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'agosto 2016. È il quarto intervento legislativo urgente, ma non si è ancora posto fine nemmeno all'emergenza. La ricostruzione sta soffocando sotto un mare di carte. Addirittura nel saldo dare-avere di questa manovrina ci sono 35 milioni in meno per quest'anno, mentre quest'anno, mentre - come tutte le altre voci - gli 885 milioni appostati nel 2018 dovranno essere confermati dalla manovra di bilancio 2018. sono due aspetti che vorrei sottolineare: il primo riguarda i *voucher* e il secondo riguarda l'allargamento dello *split payment* per i professionisti. Nell'esprimere soddisfazione per la reintroduzione del *voucher*, non possiamo però non evidenziare che, con l'approvazione di questo testo, ci troveremo di fronte a un sistema macchinoso e complesso che andrà a discapito delle famiglie. E mi riferisco alle difficoltà che incontreranno i cittadini quando dovranno registrarsi sulle piattaforme INPS. E questo non può che andare contro il nostro modo di fare politica. Il futuro del mercato del lavoro dovrà essere sempre più flessibile, ma soprattutto sempre più semplificato e snello. Siamo invece contrari all'allargamento dello *split payment* ai professionisti. Il provvedimento così formulato ha un doppio effetto negativo: quello di drenare liquidità a un settore che in questi anni di crisi è andato avanti con difficoltà e coraggio, e quello di restituire l'immagine di un Paese privo di regole certe. I professionisti oggi sono già tracciati versando la ritenuta d'acconto e l'inasprimento di regole che limitano la circolazione di liquidità è una decisione che riteniamo non produrrà reali effetti nel contrasto all'evasione. Concludendo, sarebbe necessario riflettere, in tutta onestà, su quanti errori abbia causato il rincorrere riforme istituzionali sbagliate (sto pensando alla riforma costituzionale, all'Italicum o alla riforma Delrio) e politiche economiche volte ad inseguire un momentaneo consenso (sto pensando ai vari *bonus*, ai vari interventi a pioggia a tutti i mancati tagli alla spesa improduttiva). La strada non può che essere quella coraggiosa di un taglio importante delle imposte sui redditi da lavoro e un contestuale taglio della spesa improduttiva. Ma, purtroppo, si tratta di un cammino che impone una visione pluriennale e che difficilmente una esperienza politica giunta al capolinea potrà portare a compimento. Per questi motivi, caro Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo di Forza Italia a questa ennesima fiducia.

perché questo decreto-legge è un tassello importante all'interno di una strategia di politica economica e sociale che si sta rivelando, man mano che il tempo passa, fruttuosa, perché è stata impostata in modo al tempo stesso ambizioso e concreto.

non c'è il tempo per tornare su tutti i singoli aspetti, ma i colleghi intervenuti ieri in discussione generale hanno già replicato, punto per punto: cito per tutti il collega Ichino che ha risposto, da par suo, alle obiezioni (per carità legittime, ma a nostro avviso assolutamente infondate) sulla misura a favore del lavoro occasionale. avanzate alle singole misure, ma anche e soprattutto all'impostazione generale della nostra politica economica e sociale. Ho sentito tante critiche, ma nessuno di noi è riuscito, nonostante gli sforzi nel cercare di comprendere e ascoltare le ragioni degli altri, a cogliere una strategia alternativa, altrettanto ambiziosa e ‑ mi si consenta ‑ altrettanto concreta. La strategia del Governo si è concretizzata in questi anni innanzitutto nell'obiettivo di mettere in campo politiche a favore della crescita e dell'occupazione: questo è stato il nostro principale obiettivo e lo è anche in questo decreto. Obiettivo

In termini di finalità, l'obiettivo è innanzitutto quello della crescita e dell'occupazione, ma dal punto di vista strumentale è altrettanto importante ed essenziale l'obiettivo del consolidamento fiscale e cioè la progressione verso il pareggio di bilancio e quindi la stabilizzazione del debito. Ci è stato riconosciuto da tutte le le autorità internazionali che il nostro debito è in una fase di stabilizzazione, in particolare in rapporto al PIL e naturalmente, una volta raggiunto il pareggio, l'obiettivo Il terzo importante elemento di questa strategia è mettere in campo riforme, sia dei mercati che degli apparati pubblici, finalizzate ad aumentare la crescita potenziale e la produttività complessiva del nostro sistema. In questi anni e con questo prosegue il cammino verso una riduzione strutturale della pressione fiscale e al tempo stesso una sua rimodulazione e riqualificazione.

altro che strategia delle mance e dei *bonus*, come sento continuamente ripetere! Dieci miliardi di euro di sconto fiscale ai redditi medio bassi, saldati con la riduzione dell'IMU sulla prima casa (quindi della pressione, anche in questo caso, sui ceti che posseggono la loro prima casa): due terzi di queste risorse sono andate ai consumi, quindi hanno sostenuto la crescita di questi anni. è, poi, la riduzione strutturale dell'IRAP e dell'IRES che, insieme agli incentivi agli investimenti, da quelli sulle infrastrutture edilizie a quelli sui macchinari, hanno aiutato la ripresa in atto, trainata, in particolare, dal sistema industriale. Da ultimo, le misure universali e strutturali di contrasto alla povertà. Non si tratta solo di riduzione, ma anche di riqualificazione e riorientamento della politica fiscale, proseguendo la strada della riduzione selettiva, in particolare sul lavoro e sull'impresa, finanziata anche attraverso un massiccio impegno, inedito in questa forma e in queste misure, contro l'evasione fiscale, in modo particolare contro l'evasione dell'IVA, che è la madre di tutte le evasioni*. (Applausi dal Gruppo PD*). noi vogliamo finanziare la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, sull'impresa e sulle famiglie attraverso una lotta all'evasione fiscale che ci faccia aumentare il gettito dell'IVA, non perché aumentiamo le aliquote stiamo lavorando per disinnescare le clausole che aumenterebbero le aliquote), ma perché aumentiamo il gettito attraverso misure strutturali di contrasto all'evasione fiscale. Tali misure non sono un generico impegno, ma la previsione di misure concrete. In questo decreto-legge c'è lo *split payment*, ma allo studio c'è anche l'estensione e la generalizzazione della fatturazione elettronica, che è lo strumento principe per l'eliminazione alla radice dell'evasione dell'IVA. I frutti di questa strategia stanno arrivando e lo dimostra proprio questa manovrina, che è nata per correggere uno scostamento

Come hanno riconosciuto anche le forze di opposizione, la parte forse più qualificante di questa manovrina è l'anticipo del disinnesco delle clausole dell'IVA del 2018:

che rappresenta la registrazione della conquista da parte di questo decreto-legge. È stato riconosciuto anche a livello internazionale che ci stiamo muovendo nella direzione giusta.

che il Fondo indica nell'ordine: in primo luogo, dalle politiche e dagli sforzi di riforma del Governo (questo è il primo fattore); in secondo luogo, da agevolazioni monetarie eccezionali (le politiche della Banca centrale europea, che peraltro non arrivano dal cielo, sono in gran parte anche il frutto di una politica europea del Governo italiano); in terzo luogo, dai bassi prezzi delle materie prime.

però i venti a favore diventeranno meno propizi negli anni a venire - queste istituzioni sono sempre pessimiste e preferiscono peccare di pessimismo che non di ottimismo, ed è giusto così si prevede che la crescita si attesterà all'uno per cento, quindi meno del 2017, nel 2018 e fino al 2020. Perché le previsioni sull'anno prossimo e i successivi sono più prudenti - e vorrei dire più pessimiste - rispetto a quelle dell'anno in corso? Per la fragilità finanziaria, in gran parte dovuta alla massa del nostro debito pubblico, che ci rende strutturalmente esposti a rischi; al secondo posto ci sono le incertezze politiche e al terzo le eventuali battute d'arresto al processo e al percorso di riforma.

Sgombriamo il campo dal dibattito stupido che stiamo facendo, se bisogna andare a votare un mese prima o dopo. Il problema non è la conclusione di questa legislatura, che pure è un elemento importante, ma la prospettiva: cosa succederà dopo le prossime elezioni? Avremo un Paese stabile in grado di proseguire sul percorso delle riforme o entreremo in una spirale di confusione, nella quale prevarranno gli elementi di rottura rispetto alla strada portata avanti in questi anni?

avviare una discussione che naturalmente proseguirà nel Paese e nel corpo elettorale, quando, al più tardi all'inizio del prossimo anno, saremo chiamati al voto. Quella sarà la questione decisiva. L'Europa si sta riorganizzando: ha sconfitto e isolato il focolaio d'infezione che veniva dal Regno Unito, con il rischio di una dissoluzione del percorso europeo e, in particolare, dell'Unione economica e monetaria. L'Europa va avanti, in particolare grazie al clamoroso e straordinariamente positivo risultato delle elezioni francesi: la Francia ha battuto le posizioni euroscettiche e antieuropee della signora Le Pen e ha scelto, in maniera massiccia e chiara, di restare protagonista dell'Europa e dell'euro. In Germania è scontato che il risultato a settembre sarà di continuità e stabilità, indipendentemente dal fatto che questa continuità sarà guidata dalla signora Merkel o dal *leader* della SPD Schulz. Il problema siamo noi: vogliamo essere in questo gruppo, che sta lavorando per riorganizzare, ristrutturare, riformare e rilanciare il percorso europeo dell'euro, o decidiamo di chiamarci fuori da soli? Sia chiaro che, rispetto a qualche mese fa, quando un eventuale risultato diverso in Francia avrebbe innescato una reazione a catena dissolutiva dell'Unione europea, adesso siamo in uno scenario completamente diverso. È chiaro che una crisi dell'Italia può creare danni all'Europa, ma altrettanto lo è che gli altri Paesi hanno deciso di andare avanti. Il problema è nostro: vogliamo essere dentro questa discussione da protagonisti o vogliamo ritagliarci uno spazio di fuga che ci porterebbe - questo sì - a una condizione d'instabilità pericolosa e di recessione? Questo credo sia il tema politico che è davanti a noi. Il Governo - e il Partito Democratico che lo sostiene, insieme all'apporto determinante di altri alleati è chiaramente orientato verso questa direzione: siamo per far andare avanti l'Europa e partecipare alla discussione e alla progettazione di una fase nuova per l'Europa e per l'eurozona in particolare. Per questa ragione, votiamo la fiducia a questo Governo

Signor Presidente, non voterò la fiducia al Governo in dissenso dal Gruppo che mi ospita, soprattutto per segnalare una vicenda di cattiva politica: quella dei *voucher* e della regolazione che li sostituisce. Se è ben vero che la società chiede regole semplici, certe e stabili per orientarsi all'attività, nel corso di questa legislatura la disciplina relativa ai lavori brevi è cambiata addirittura quattro volte. Prima è stata ampliata rispetto al precedente sedimento normativo, poi è stata corretta con l'opportuna introduzione di adempimenti funzionali alla vigilanza, successivamente è stata cancellata di fronte alla minaccia referendaria, infine è stata reintrodotta in termini che scontentano tanto l'ideologia quanto la realtà. Il nuovo testo viene introdotto non solo dopo la fuga dal confronto referendario, ma con modalità che non ne consentono, di fatto, un'attenta lettura parlamentare, e si vede. Si riconosce l'esigenza di regole semplici del lavoro breve, ma la si soddisfa evocando la pesante disciplina del lavoro subordinato e, inspiegabilmente, solo nelle imprese fino a cinque addetti, come se la realtà fosse fatta per segmenti. L'unico limite importante - quello dei compensi tra lo stesso committente e lo steso lavoratore - è perfino troppo generoso, ma poi si aggiungono limiti ingiustificati ai compensi tra un committente e più prestatori e tra un prestatore e più committenti. I contratti di lavoro intermittente restano inibiti da vincoli senza senso e tutto questo risvegliando inutilmente pregiudizi ideologici. Gente di Governo, meditate sul fatto che avete scontentato tanto chi idealizza il lavoro, quanto coloro che il lavoro lo fanno. Non mi sembra, però, che i tanti scontenti diano luogo a tanto onore.

noi teniamo alla legittimità della rappresentanza parlamentare e alla regolarità dei voti. Stiamo votando una fiducia importante e altre fiducie importanti sono programmate per le prossime settimane. sappiamo che alcuni colleghi sono stati eletti sindaci in città con più di 20.000 abitanti. Sappiamo che c'è un'incompatibilità tra le due cariche, che prevede un *iter* abbastanza lungo

nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge, con modificazioni,

Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini,

Rizzotti, Romani Paolo,

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge, con modificazioni,

Tale provvedimento è arrivato in Commissione nell'ottobre 2015, quindi giace in quella sede da un anno e otto mesi.

Perché? Noi abbiamo presentato 8.000 emendamenti e in passato ne ho presentati 85 milioni, ma quando si è voluto fare una legge, la si è fatta:

perché ci sono i ballottaggi, ma bisogna dare anche il contentino a sinistra, quindi, non per un pugno di dollari ma per un pugno di voti, si sta svendendo la nostra identità; si sta svendendo l'identità dei cittadini italiani.

il numero delle cittadinanze rilasciate al livello europeo sta regolarmente calando. Qual è il Paese che nel 2016 ha fatto il *record* del numero di cittadinanze rilasciate? L'Italia con

Dirò di più: il signore di Manchester, figlio di libici che grazie allo *ius soli*, cioè quella legge che oggi volete portare avanti, ha preso la cittadinanza e il passaporto inglese, ha fatto l'attentato a Manchester e, *dulcis in fundo*, aveva preso 7.500 euro di borsa di studio e invece di studiare con quei soldi ci ha comprato la bomba. Bravi, complimenti! *(Applausi dal

Qualcuno ha detto che siamo pronti a metterci la fiducia. Abbiamo qui il ministro Finocchiaro, siamo già pronti, mettiamola già oggi, senza neanche la discussione generale, ma ricordatevi che con una fiducia non si fa niente, dovesse essere approvato con un voto di fiducia, un articolo interamente sostitutivo, poi tornerebbe alla Camera e là morirebbe. Oppure preparatevi a metterne quattro. Vi auguro buona fortuna e buon voto a tutti.

una precisazione, Presidente. Questa è la dimostrazione di cosa state facendo. Voi state consegnando il dibattito... voi state consegnando il dibattito su un tema così importante a queste esternazioni, da cui mi dissocio, e ad altre che sentirò

di conseguenza abbiamo l'obbligo di farlo adesso. C'è la possibilità di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, ma non quando si rischia, a causa di questo, di venire meno ad un preciso obbligo previsto dal Regolamento. In secondo luogo, la mia obiezione è che quest'anticipazione viene fatta non solo contro il Regolamento, ma contro la Costituzione, che all'articolo 72, comma 1, prevede che ogni disegno di legge sia esaminato dalla Commissione e dall'Assemblea.

Tanto meno si può anticipare un provvedimento non discusso in Commissione a danno di un punto che l'ordine del giorno ed il Regolamento prescrivono tassativamente: non è che si poteva fare oggi, ma possiamo farlo tra due o tre settimane come una mozione qualsiasi.

sottoposti alle Camere entro cinque giorni dalla loro emanazione. Questo, pertanto, è un termine fondamentale. Se il Parlamento decidesse che non ci sono i presupposti, il decreto-legge decadrebbe. È un obbligo costituzionale, non è uno dei uno dei tanti punti, con tutto il rispetto per ciascun punto del Regolamento. È un punto fondamentale che non possiamo rinviare. Si esamina questo e poi si deve andare avanti con l'ordine del giorno normale.

ove ne faccia richiesta entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato e su questo viene fatta una votazione nominale con scrutinio simultaneo.

mi ha fornito gli argomenti che motivano questo nostro voto e lo ha fatto quando ha ricordato il numero degli emendamenti presentati in Commissione, che sono la ragione

questo brevissimo dibattito che ha preceduto il mio intervento mi conferma sempre l'esistenza di un atteggiamento ostruzionistico nei confronti di questo testo. altresì dirvi con molta franchezza una mia opinione personale. Naturalmente tutte le condotte parlamentari previste dal Regolamento sono legittime, ma credo che politicamente non sia un atto nobile da parte del Parlamento quando, invece di discutere nel merito, si abbandona

dall'intervento del senatore Calderoli ho capito che esiste un problema ulteriore, relativo cioè alla necessità che noi si discuta di questo disegno di legge dopo averlo letto, perché senza averlo fatto le questioni diventano più complicate. Noi non stiamo parlando soltanto di dare la cittadinanza a dei bambini e a dei ragazzi che sono nati in Italia,

Io mi auguro che il dibattito in Assemblea su questo provvedimento non abbia a seguire la linea ostruzionistica che è stata invece invece introdotta in Commissione e sia veramente un dibattito importante nel merito del disegno di legge. MALAN

Presidente).* Senatore Volpi, questo stigmatizza il suo stile da senatore.

è affrontata la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto *ius e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto *ius culturae*. Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 e, una volta trasmesso al Senato, è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, che ne ha iniziato l'esame il 27 ottobre 2015, con la relazione introduttiva della relatrice Lo Moro. Dopo la discussione e la reiezione delle questioni pregiudiziali proposte da alcuni Gruppi di opposizione,

finestra"). L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 2856: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,

per cortesia. Nel corso della seduta del 14 giugno scorso la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di

Presidente, prima di intervenire sul merito, faccio un richiamo al Regolamento. Lei ha completamente disatteso quanto previsto dal nostro Regolamento, perché ha espulso dall'Aula

di ristabilire l'ordine, sospendendo la seduta e concedendomi di poter prendere la parola tranquillamente, non obbligando il presidente Torrisi a consegnare un testo scritto, perché gli è stato impedito di parlare, così come avvenuto al senatore Mancuso. Presidente, le chiedo di applicare il Regolamento. Quando verrà applicato, prenderò la parola. PRESIDENTE. Senatore Calderoli, abbiamo proceduto comunque dopo che era stata data la parola al senatore Torrisi per l'illustrazione.

Si prevede l'impossibilità di accedere agli asili nido o alle scuole materne per coloro che non hanno eseguito le vaccinazioni; a livello della scuola dell'obbligo, è invece prevista una sanzione da 500 a 7.500 euro ed, eventualmente, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, in particolar modo, al tribunale dei minori. Presidente, sono adulto, addirittura un po' vecchio, sono vaccinato e sarei fuorilegge in questo momento: ho fatto vaccinare mio figlio e credo fortemente nei vaccini e nei loro effetti benefici.

Il relatore nel corso della discussione in Commissione mi ha detto che quello che vale in Lombardia può non valere nel resto del Paese, citando le parti meridionali dove, a suo avviso, non esiste ancora una cultura vicina alla vaccinazione, facendo al contempo il parallelo con la cultura della donazione degli organi. La cosa mi ha stupito perché dopo aver visto con sorpresa un Governo intervenire con un decreto-legge su una questione come quella delle vaccinazioni, non vorrei, senatore Mancuso, trovarmi la prossima volta un decreto-legge che obblighi a donare gli organi e lo Stato che fa una specie di magazzino con tanti fegati e cuori, per poterli usare come merce di ricambio.

grandissimi risultati: l'informazione, la consapevolezza e il diritto di poter liberamente decidere. Questi sono i presupposti che a mio avviso devono essere applicati. Rispetto al fatto che siano o no sussistenti i presupposti di necessità e urgenza,

ha affermato che non si ha, al momento, una situazione di emergenza nazionale; appare pertanto di tutta evidenza che non sussistono i presupposti fattuali per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non solo.

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

vada ad introdurre non il divieto di ingresso, ma il pagamento da 500 a 7.500 euro di multa. Allora cosa c'è? Il ricco va a scuola e ogni anno paga e il poveretto invece resta fuori?

saputo mettere dei paletti economici rispetto ad un diritto-dovere che è un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale. Proseguiamo con il secondo che, tra l'altro, consente - e ci sarà modo di divertirsi - il voto segreto. Tale comma stabilisce: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». E mi viene ancora più da ridere se penso che quelli che non pagano e non vaccinano il bambino possono vedersi segnalati dalla ASL al tribunale dei minori e vedersi, sotto la discrezionalità del giudice, revocata la patria potestà del proprio figlio. È rispetto della persona umana togliere un bambino alla propria famiglia? Proseguiamo:

ricorso. Ma più che agli articoli della Costituzione, credo che questo provvedimento sia contrario al buon senso. Non è con le grida manzoniane o con gli obblighi di legge che si sensibilizza una persona a farsi vaccinare. Bisogna istruirla, formarla, renderla consapevole e poi andrà a vaccinarsi spontaneamente. Io dico sì ai vaccini, ma no agli obblighi. Informiamo i genitori, facciamo loro sapere attraverso i medici di famiglia quali sono i vantaggi possibili e i rischi di una vaccinazione, ma poi ciascuno decida a casa Con questo decreto-legge otterrete l'effetto opposto. Si sta risvegliando una curiosità e una diffidenza da parte delle famiglie, per cui al posto di vedere aumentare il tasso di vaccinazione, lo vedrete decrescere.

ho la sensazione che lei, non di rado, trascuri chi da questa parte dell'emiciclo le chiede la parola. Credo che le abbia una considerazione di senatori

Mi faccia finire, la prego. Come dicevo, non ho ascoltato la relazione del relatore. Lei ha detto che sarà depositata. Nel momento in cui ha incardinato quel provvedimento, in quest'Aula non si capiva che cosa stesse accadendo: i banchi del Governo e lei, nonostante ciò, ha ritenuto di raggiungere lo scopo di un incardinamento che non fa bene a quel provvedimento.

sull'obbligo delle vaccinazioni, a mio avviso, non ci sono assolutamente problemi di costituzionalità, perché la tutela della salute è anche tutela dei terzi, oltre che diritto alla cura.

Non mi preoccuperei, invece, per quanto è stato detto da certe campagne antivacciniste in merito agli eventi avversi da vaccinazione.

nascono circa 500.000 bambini all'anno, quindi posso attendermi un effetto avverso da vaccinazione ogni sei anni. Contemporaneamente, invece, per quanto riguarda il morbillo, si possono avere anche mille morti, come si è verificato - nel mondo vaccinato, tra l'altro tra l'altro - nell'ultimo anno (poi le cifre possono variare). Quindi, un effetto avverso ogni 3 milioni è sicuramente preferibile a mille morti in un anno.

urgentemente l'obbligo, entro settembre, perché non siamo preparati a farlo. Da questo punto di vista, come dice lei, il discorso entra nel merito del decreto-legge emanato e delle proposte emendative. Per me si può tranquillamente

Signor Presidente, avremmo tempo e modo di discutere nel merito di questo decreto-legge. Arrivo subito al dunque. Per quanto ci riguarda, confermiamo il nostro voto contrario, che abbiamo

Presidente, prima di entrare nella questione dei presupposti costituzionali sul decreto-legge in materia di vaccini, va chiarita la valenza del dibattito: stiamo discutendo non dell'utilità dei vaccini, ma di come il Governo interviene su una materia tanto delicata. Il Movimento 5 Stelle ha elaborato le sue proposte per un sistema vaccinale moderno, basato su evidenze scientifiche e in linea con le migliori pratiche dei Paesi più avanzati. *(Commenti ha "calato" invece un provvedimento normativo che la Costituzione ammette solo in limitate ed eccezionali condizioni. Siamo qui a discutere della costituzionalità di questo strumento. I decreti-legge traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati a operare immediatamente, per fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007, ha rilevato come non sia sufficiente che la necessità e l'urgenza siano apoditticamente enunciate, bensì rileva l'effettivo e concreto bisogno di un intervento normativo urgente: insomma, ci deve essere un'epidemia o un rischio conclamato di epidemia. L'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di 12 tipi di vaccinazioni, triplicando il numero di vaccini obbligatori previsti attualmente. A questo proposito va rilevato che i requisiti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione, che in questa sede rilevano, dovrebbero, pertanto, avvincere l'intero ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico complessivo, concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare. Dovremmo cioè avere 12 emergenze in atto. Dovremmo pensare che l'intero sistema di sorveglianza epidemiologica nel nostro Paese sia saltato e dovreste chiedere voi, innanzitutto, le immediate dimissioni del ministro Lorenzin. La cogenza di un'epidemia in corso (o, più precisamente, di più epidemie in corso) è, però, confutata dallo stesso piano vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute che, nel gennaio 2017, non evidenziava alcun tipo di emergenza, né di epidemia. Si può obiettare che il piano risale al lontano mese di gennaio, lo stesso Presidente del Consiglio, all'atto della presentazione del decreto-legge in oggetto, ha dichiarato che non sussiste alcuna emergenza nazionale. Dunque, la necessità e l'urgenza di un simile decreto è un'invenzione e lo dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, lo stesso *iter* di approvazione del decreto-legge, a dir poco ridicolo. Ricordo in proposito alcune date. Giovedì 11 maggio la ministra Lorenzin annuncia un decreto-legge sui vaccini lo stesso 11 maggio interviene formalmente il Governo precisando che l'indomani non ci sarebbe stato alcun decreto-legge sui vaccini all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Venerdì 12 maggio il Consiglio dei ministri esamina una bozza del decreto-legge. Venerdì il 19 maggio, dopo una settimana, il Consiglio dei ministri approva il decreto-legge, ma il testo rimane fantasma e scoppiano polemiche interne al Governo, con il ministro Fedeli che contesta la violazione del diritto allo studio.

perché aspettare diciotto giorni, nei quali potrebbero morire o infettarsi migliaia di persone? Più credibile è che il tempo sia occorso per trattative interne e coprire, ma non del tutto, le pudenda del Governo. A questo punto è chiaro che le necessità e l'urgenza sono ipotesi fantasiose, e più fondato sarebbe, allora, chiedere le dimissioni dell'intero Consiglio dei ministri per procurato allarme. Ma non è tutto. Connesso ai presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione è il criterio di ragionevolezza, legato a sua volta a quello della proporzionalità. Introdurre l'obbligatorietà vaccinale per una quantità abnorme di vaccini non c'è un caso simile in tutta Europa - attraverso la decretazione d'urgenza contrasta, infatti, in maniera diretta e indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione. La previsione di dodici trattamenti vaccinali obbligatori non risulta proporzionato né al risultato annunciato, né al fine perseguito dal legislatore. Peraltro i presupposti costituzionali per la emanazione

la decretazione d'urgenza contrasta in maniera diretta e indiretta anche con il principio di ragionevolezza. In relazione all'articolo 32 della Costituzione, ricordo che «nessuno può essere obbligato la legge è vincolata in questo senso, perché in nessun caso possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana». E una misura che comprima la libertà imponendo obbligo di cura dovrebbe essere certa, ordinaria, stabile, condivisa, direttamente approvata dal Parlamento e non un decreto-legge che, per sua natura, è provvisorio. L'adozione di un simile provvedimento in vista del nuovo anno scolastico fa scattare un obbligo in capo alle famiglie. Scuole materne e asili si apprestano a chiedere le certificazioni delle vaccinazioni; avremo famiglie costrette a vaccinare senza garanzia che il decreto-legge convertito (ovvero in che forma sarà convertito), pena il diniego di iscrizione. Già la sanzione è irragionevole: ammesso e non concesso che rifiutare dodici vaccinazioni in blocco costituisca omessa tutela per un minore e non, invece, la protezione da un evento stressante per un sistema immunitario immaturo, è assurda una sanzione che ricade proprio sui bambini e li priva del diritto di frequentare asili e scuole materne. Né si può addurre in modo generico e superficiale la difesa del diritto alla salute per gli altri bambini, su vaccinazioni che hanno risibile rilevanza nell'infanzia (epatite B) o alcun rischio infettivo (antitetanica).

Ed è il Governo stesso a palesare il costrutto incongruo, laddove fa scattare il divieto di iscrizione per le scuole materne e non per le scuole elementari o medie, come se il Governo ritenesse - e mi riferisco all'epatite B - più probabile lo scambio di siringhe, le trasfusioni in classe o i rapporti sessuali tra bambini rispetto ai preadolescenti. *(Commenti Vergognatevi. Siete voi che create questo paradosso, e non io che lo denuncio.

In più punti appaiono violazioni dei presupposti di necessità e urgenza, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità connessi. È evidente che si sta abusando dello strumento della decretazione e su questo abbiamo espresso in Commissione affari costituzionali il nostro voto contrario. Abbiamo portato in quest'Aula il dibattito perché sia chiaro davanti agli italiani come il Governo interviene su materie delicatissime come la salute, il diritto e la libertà di cura, la famiglia, la tutela dei minori, il diritto alla salute e all'istruzione. Il dibattito va sottratto agli appetiti propagandistici del Governo e affrontato con responsabilità, rigore giuridico e scientifico. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Il Movimento 5 Stelle - ripeto - ha già elaborato le sue proposte per un sistema di vaccinazioni moderno, Le abbiamo lette! ENDRIZZI *(M5S)*. E chiama il Governo e la maggioranza a un confronto parlamentare serio e non frettoloso, come vorreste. Per questo esprime voto contrario alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Presidente, io porto un grande rispetto per il suo ruolo istituzionale e, ovviamente, per la sua persona. Non sono, però, disponibile - e credo come me molti altri colleghi - a ignorare che sono stati varati alcuni precedenti, pochi minuti fa,

la sua meraviglia nel registrare un atteggiamento a dir poco confidenziale del collega Volpi nei suoi confronti che l'ha amareggiata. Ancor più meraviglioso è il principio in base al quale lei, che è il Presidente del Senato e al quale non devo insegnare nulla,

Non è poi comprensibile quale articolo del Regolamento consenta

la profilassi vaccinale uno strumento utile e indispensabile per la salute dei cittadini. Tuttavia, qui non stiamo discutendo se i vaccini come lei ha giustamente sottolineato durante l'intervento di un altro collega, ma stiamo discutendo se sussistano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione per un decreto-legge su questo argomento. Il Presidente del Consiglio ha detto di no,

Esiste al mondo una statistica su 12 vaccinazioni obbligatorie? Non esiste, perché non c'è alcun Paese al mondo che imponga 12 vaccinazioni obbligatorie.

che fare personalmente. Ci sono centinaia, migliaia di medici, molti dei quali pediatri, che non consigliano, anzi sconsigliano la vaccinazione contro la varicella.

prevede che le famiglie impongano ai loro figli un numero di vaccini più alto di qualunque altro Paese al mondo.

incredibile che non dovrebbe avere nessuno, quello di portare via i bambini ai loro genitori. Ci sono poi altre incongruenze nel decreto-legge. C'è l'obbligatorietà assoluta assoluta per istituzioni del tutto facoltative come l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, mentre c'è un'obbligatorietà mitigata per la scuola dell'obbligo.

Stavo dicendo che qui non stiamo discutendo dell'obbligatorietà della scuola, per cui non c'è bisogno di un decreto. Stiamo discutendo di un fatto di salute. Se si tratta di un fatto di salute, bisognerebbe studiarlo meglio e scrivere qualcosa che non sia palesemente illogico.

incardinato, si fanno venire in Italia, prelevandoli direttamente dalle coste africane, centinaia di migliaia di persone le quali - secondo le statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità - sono ad alto o altissimo rischio

era quando si sacrificavano i primogeniti agli idoli! Questo è l'idolo dello Stato e io non voglio sacrificare neanche un'unghia di un bambino!